il senatore Pedica

il costo medio mensile delle malattie rare, per le famiglie che si trovano a far fronte a queste patologie, supera i 500 euro, almeno nel caso di una famiglia su quattro, e può arrivare oltre i 2.000 euro. Dall'indagine emerge che le famiglie sotto la soglia di povertà sono più numerose della media italiana stimata dall'ISTAT nel 2009. Se a queste si aggiungono le famiglie che possono essere considerate a forte rischio di povertà, si arriva ad una percentuale del 35 per cento. Almeno il 20 per cento delle famiglie intervistate ha dovuto ricorrere ad un aiuto finanziario che, per più della metà dei casi, è stato fortunatamente offerto dai parenti. Signora Sottosegretario, come lei certamente saprà, i costi di assistenza e cura per le malattie rare, in termini di aiuto umano e tecnico, sono molto elevati, così come alti alti sono quelli dei pochi farmaci esistenti. Mi riferisco, in particolare, ai farmaci orfani, così definiti perché le industrie farmaceutiche ne trascurano sviluppo e commercializzazione proprio in quanto prodotti destinati al trattamento di un ristretto numero di pazienti, e quindi e quindi poco allettanti economicamente. Tra l'altro, ed il dato è grave, gran parte dei malati afflitti da queste patologie sono invisibili per il sistema sanitario nazionale, a causa del mancato inserimento di oltre un centinaio di malattie rare nell'allegato A del decreto ministeriale n. 279 del 2001, che contiene, come è noto, un elenco corrispondente comunque ad una piccola parte delle oltre 6.000 malattie rare ad oggi scoperte. Secondo una stima, nel 2004 il numero degli italiani affetti da malattie rare era pari a 1,5 milioni. Signora Sottosegretario, purtroppo pare che tale stima, già molto elevata, sia ulteriormente salita e che spesso si tratti di pazienti in gran parte sconosciuti alla sanità pubblica. La situazione è molto preoccupante, soprattutto se pensiamo che in gioco vi è uno dei beni più importanti per il Paese, il diritto alla salute di tutti i cittadini, costituzionalmente garantito dall'articolo 32 della nostra Carta. Per questi motivi, sottolineando ancora una volta la primaria rilevanza del bene salute, chiedo al Governo se abbia intenzione di predisporre ed avviare un programma nazionale triennale sulle malattie rare, malattie rare, di istituire un fondo nazionale per le malattie rare, che garantisca la ricerca e lo sviluppo dei farmaci orfani e l'accesso ad essi per i pazienti, affidando compiti consuntivi e propositivi sulla gestione del fondo a un comitato nazionale per le malattie rare da malattie rare. Chiedo inoltre al Governo se ritenga che la defiscalizzazione della ricerca sui farmaci orfani possa incentivare le case farmaceutiche alla loro produzione e quindi se si voglia considerarla come un'iniziativa utile e perseguibile. PRESIDENTE. La della salute, e di attivarsi al fine di ottenere la disponibilità e la gratuità dei farmaci, dei dispositivi medici e di quanto sia utile per la cura ed il trattamento dei pazienti afflitti da malattie rare. Chiedo

rare, ricordo che il legislatore, con la legge n. 326 del 2003, che ha istituito l'AIFA, ha disposto che il 50 per cento del Fondo istituito presso la stessa Agenzia, attraverso un apposito contributo del 5 per cento delle spese autocertificate versato dalle aziende farmaceutiche, sia destinato alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego di farmaci orfani per le malattie rare e di medicinali che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie. Per quanto attiene alla defiscalizzazione della ricerca sui farmaci orfani, si ritiene che promuovere e facilitare lo sviluppo e la ricerca sui farmaci orfani risponda ad un'esigenza etica per cui l'impegno economico per la commercializzazione degli stessi, essendo importante e rischioso, deve essere incoraggiato da leggi specifiche. In tal senso sono state intraprese iniziative sia a livello nazionale che europeo dalle autorità della salute, al fine di offrire gli incentivi necessari per incoraggiare da una parte lo sviluppo dei farmaci orfani, dall'altra l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione attraverso una procedura centralizzata. In merito alla disponibilità e gratuità dei farmaci e dei dispositivi medici per i pazienti affetti da malattie rare, evidenzio che in Italia la normativa consente già il pagamento delle cure dei malati affetti da malattie rare da parte del Servizio sanitario nazionale. Per i pazienti affetti da malattie rare è prevista, sulla base del decreto del Ministero della sanità n. 279 del 18 maggio 2001, l'esenzione dal pagamento della quota fissa per le prestazioni farmaceutiche e specialistiche. Parallelamente le Regioni, sulla base del fabbisogno della propria popolazione, possono predisporre modalità di acquisizione e di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici, anche mediante la fornitura diretta da parte dei servizi farmaceutici pubblici. In alcune Regioni, pur non essendovi alcuna normativa regionale che disciplini l'erogazione di farmaci destinati alla cura di pazienti affetti da malattie rare, è prassi consolidata autorizzare tale fornitura, su richiesta specifica delle aziende sanitarie e previa valutazione della relativa appropriatezza terapeutica, tenuto conto dei protocolli clinici concordati dai presidi della rete con il centro interregionale di riferimento per le malattie rare. Riguardo alla possibilità di usufruire, a carico del Servizio sanitario nazionale, di farmaci (anche se di fascia C) necessari alla terapia e al trattamento sintomatico di malattie rare, autorizzati per indicazioni terapeutiche diverse da quelle di interesse, osservo che questi farmaci possono venire somministrati nel corso di trattamenti eseguiti in regime di *day hospital* per consentire ai soggetti affetti da tale malattia di usufruirne senza sostenerne il costo. Infatti, nei casi in cui sia deciso che possa rendersi indispensabile per il trattamento di singoli pazienti, il farmaco potrà essere utilizzato con indicazione personalizzata sotto la diretta responsabilità del medico prescrittore,

in base alla quale il trattamento con specialità medicinali registrate per altre indicazioni terapeutiche, in una struttura pubblica o privata accreditata su paziente ricoverato, (anche in regime di *day hospital*) è comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, essendo la tariffa di ricovero comprensiva anche del trattamento farmacologico praticato. Concludendo, osservo che l'insieme delle azioni intraprese negli anni da parte del Ministero della Salute e dalle Regioni si configurano già come una strategia piuttosto avanzata a sostegno delle malattie rare, soprattutto se confrontata con quelle di altri Stati europei, e che il Ministero della Salute è favorevole a predisporre un Piano nazionale per le malattie rare ed opererà dunque in questo senso.

Quindi richiamerei il Governo a mantenere questo impegno. In più, non è così vero che tutti i pazienti affetti da malattie rare hanno il rimborso gratuito: dipende molto dalle Regioni, sottoposte anche a piani di rientro. Per esempio, ci sono patologie che usano farmaci cosiddetti *off label*, presenti in fascia C, C, che non sono rimborsabili. Sono pazienti affetti da malattie rare, tipo la malattia di Leber, che è una neuropatia ottica, che devono sborsare cifre considerevoli per il trattamento della patologia. che non tutte le ASL si comportano allo stesso modo, non tutte le Regioni si comportano allo stesso modo, sostanzialmente abbiamo disuguaglianze fra i pazienti affetti da malattie rare sul territorio nazionale: non sono tutti trattati nello stesso modo, e questo è comunque anticostituzionale, oltre che chiaramente contrario alla dignità del malato. Io penso che Parlamento e Governo debbano farsi carico di rendere omogenee sul territorio nazionale le cure - per questo forse servirebbe un disegno di legge porre anche rimedio ad alcune ingiustizie per cui alcuni farmaci di fascia C sono erogati per malattie rare in alcune ASL, ma non in altre. Oltretutto, c'è un'enorme complicazione a carico dei pazienti per riuscire a svolgere tutte le pratiche per arrivare alla definizione dell'eventuale gratuità del rimborso, che deve essere per di più rinnovato

Ringrazio il Governo per la spiegazione che, come per il collega che mi ha preceduto, non mi ha soddisfatto al

al fine di fornire informazioni in merito allo stato delle domande di adesione presentate dai soggetti danneggiati, di cui si fa cenno appunto nell'interrogazione, faccio presente che è stata appositamente creata, sul sito istituzionale del Ministero della salute una sezione speciale sul tema delle transazioni, già attiva a partire dalla fine dell'anno 2009, per consentire ai legali di parte di presentare le domande di adesione attraverso la piattaforma informatica realizzata. La stessa sezione è stata più volte utilizzata per pubblicare avvisi e comunicazioni sull'argomento. L'ultimo avviso è stato pubblicato lo scorso 2 marzo: sono stati forniti elementi informativi sull'*iter* della bozza di decreto interministeriale per la definizione dei moduli transattivi da corrispondere ai soggetti che hanno presentato domanda di transazione, come previsto dal decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132, ed è stata ripristinata la linea telefonica dedicata al pubblico, attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 13, al numero 06 59943135, per informare i diretti interessati sullo stato delle pratiche. Rispetto al contenuto degli altri quesiti formulati, il Ministero sta seguendo la procedura transattiva prevista e disciplinata dalle disposizioni normative vigenti, sia per ciò che attiene la relativa programmazione economica che per gli aspetti connessi alla gestione dell'intera procedura transattiva che, come è noto, si perfeziona con un decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato. Al riguardo preciso che la procedura per l'adozione del provvedimento è in fase avanzata, in quanto si è già al secondo confronto con l'Avvocatura generale dello Stato. Da ultimo, il Ministero della salute indica la posizione favorevole circa ogni ulteriore iniziativa normativa idonea a garantire la piena soddisfazione dei soggetti interessati alla tematica sollevata dall'interrogazione in esame.

quello degli emotrasfusi è un problema annoso - come sappiamo - per il Parlamento italiano, per il Governo, e riguarda un numero di pazienti, se vogliamo, non enorme, ma sicuramente colpiti da una situazione di sofferenza molto particolare,

insufficiente a far fronte a tutte le necessità che ci sono e anche ai nuovi bisogni che emergono (e per i quali tante volte anche questo Parlamento si è impegnato con risposte negative da parte del Governo, anche nelle ultime leggi in ci sembrava giusto garantire ai pazienti che hanno aderito alla transazione almeno la facilità dell'accesso e dell'informazione e anche tempi congrui per l'erogazione della cifra stabilita dalla transazione Purtroppo, invece, questi pazienti stanno aspettando da anni e, nonostante gli sforzi che il Sottosegretario adesso ci ha illustrato, l'informazione è assolutamente carente,

e quando si accede le risposte talvolta sono sconfortanti, non sono esaustive, non viene data una risposta precisa al paziente, del tipo: «La sua pratica è la n. 150 e verrà erogata fra un mese e mezzo».

senza magari dover telefonare, sottoporsi a ore di attesa al telefono e magari a qualche risposta scortese; oltretutto si richiedeva di sollecitare (questo l'ho fatto più volte personalmente al Ministro, e lo faccio ancora) ancora) la velocità con cui queste pratiche transattive possono essere liquidate. Quindi, si chiede velocità nella liquidazione (perché mi pare che ormai il lavoro dell'ufficio sia avviato: si tratta solo, appunto, di svolgere le pratiche) e informazione al paziente. Penso che non costi veramente nulla attribuire al paziente un codice con cui possa accedere, visto che c'è già la pagina *web*,

esaurire la propria esperienza terrena, che speriamo sia la più lunga possibile; ma purtroppo sono già successi questi casi e non ci sembra giusto da parte dello Stato rispondere in questo modo ai cittadini più sfortunati.

quanto segue circa il concorso a 145 posti di dirigente tecnico indetto dal Ministero in data 30 gennaio 2008. In via preliminare, ritengo opportuno evidenziare che il Ministero, nel predisporre il bando di concorso, si è scrupolosamente attenuto alle indicazioni e ai principi espressi dal Consiglio di Stato, con parere n. 6148 del 3 novembre 2007, a tal fine espressamente richiesto. Specificamente, i criteri posti a fondamento del bando hanno tenuto conto della funzione fondamentale del dirigente tecnico presso il Ministero, il quale ha pertanto ritenuto necessario, nell'ambito del sistema generale di reclutamento delineato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, individuare elementi di compatibilità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 1994 che rimane, comunque, la norma più idonea a garantire la specificità della figura professionale del dirigente tecnico medesimo. Sicché, sulla base di questa impostazione, l'amministrazione ha stabilito quali dovevano essere le norme da cui desumere i destinatari del bando, i requisiti e le modalità di partecipazione, la composizione delle commissioni e il regime delle prove d'esame. In particolare, l'articolo 6 del bando ha previsto che l'esame, articolato in tre prove scritte e una orale, è preceduto da prove preselettive consistenti in una serie di quesiti a risposta multipla e che viene ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ogni settore o sottosettore. Come è noto, per effetto della partecipazione di numerosi candidati a più settori, si è verificato che molti di loro sono stati ammessi a partecipare alle prove scritte per più di un settore e, conseguentemente, il numero degli ammessi è stato pari a 1477, comprensivi di candidati presenti in più settori. Alcuni candidati hanno impugnato dapprima l'esclusione dalle suddette prove scritte e, successivamente, il provvedimento con il quale il Ministero, nel dare esecuzione alle ordinanze cautelari adottate dal TAR per il Lazio sui ricorsi proposti dai ricorrenti medesimi, li aveva nuovamente esclusi dalle prove scritte del suddetto concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico. Il Ministero si è trovato, infatti, nella delicata situazione di dover individuare le condizioni e i limiti imposti dalle ordinanze di sospensiva del TAR del Lazio. L'Amministrazione ha quindi proceduto alla compilazione di un elenco di candidati formato sulla base del punteggio conseguito nella prova preselettiva prescindendo dai settori disciplinari, fino al raggiungimento della posizione n. n. 1.450, corrispondente al punteggio di 24,50. La compilazione di tale elenco, tuttavia, non avendo alcuna valenza formale, non è stata pubblicata ma soltanto comunicata ai ricorrenti interessati attraverso i loro legali. Essa è stata soltanto lo strumento tecnico-operativo con il quale è stata ricostruita la teorica ed astratta graduatoria che individuava il limite massimo dei 1.450 nominativi, stabilito in via generale, dall'organo giudicante con i provvedimenti cautelari adottati. È evidente, però, conformemente ai principi regolanti gli effetti del giudicato amministrativo, che le ordinanze del TAR del Lazio relative alle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti di esclusione dei candidati dalle prove scritte, non possono in alcun modo giovare a coloro i quali non hanno ritenuto di proporre ricorso, stante, nei confronti dei soggetti che hanno fatto acquiescenza, l'espresso divieto legislativo dell'estensione del giudicato medesimo. Infatti, l'attuazione delle suddette ordinanze ha prodotto i propri effetti limitatamente a quei candidati che, avendo presentato ricorso avverso l'esclusione dalle prove scritte con contestuale istanza di sospensione

Il suddetto *modus operandi* dell'Amministrazione è stato, peraltro, dichiarato legittimo sia dal costante orientamento del TAR del Lazio, sia dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il quale, decidendo su tutti i ricorsi presentati in appello dai candidati esclusi, ha confermato che l'amministrazione aveva dato puntuale esecuzione alle ordinanze cautelari del TAR del Lazio, respingendo gli appelli medesimi. L'esattezza della modalità di esecuzione da parte dell'amministrazione, al contrario di quanto affermato nell'interrogazione, è stata pienamente avvalorata e confermata anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva, il quale ha finora espresso un uniforme e costante parere di reiezione nei confronti dei candidati esclusi che hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato. predetti pareri l'organo consultivo, decidendo nel merito dei gravami in questione e assorbendo le eventuali precedenti pronunce cautelari, testualmente ha argomentato che il bando del concorso in esame ha stabilito che sarebbe stato ammesso un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ogni settore o sottosettore. I ricorsi si fondano sull'implicita premessa che dovessero essere ammessi complessivamente 1.450 candidati; tale tesi non è suffragata da nulla, perché in nessuna parte del bando è stabilito che dovessero essere ammessi agli scritti complessivamente 1.450 candidati.

essa sarebbe stata esposta alle fondate impugnazioni dei concorrenti risultati idonei non vincitori nelle graduatorie finali; perché è evidente che, col sistema propugnato dai ricorrenti, potrebbe essere ammesso alle prove un numero di concorrenti superiore al decuplo del settore o sottosettore considerato, violando così la disposizione del bando e vanificando lo scopo della preselezione. Per le considerazioni sopra esposte non si ravvisano i presupposti e le motivazioni per dar luogo ad eventuali prove suppletive per i candidati che, pur rientrando tra i primi 1.477 del suddetto elenco, non sono stati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso in questione, così come richiesto nell'interrogazione. Le prove scritte si sono concluse il 24 marzo scorso ed è attualmente in corso l'esame degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle stesse prove.

Signora Presidente, l'Arma dei carabinieri ha sviluppato un graduale processo di rinnovamento e di razionalizzazione ed è in tale contesto che devono inquadrarsi tutte le iniziative di ordinamento strutturale realizzate al fine di corrispondere, con sempre maggiore efficacia, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per far fronte ai nuovi compiti attribuiti all'istituzione, quale forza di polizia ad ordinamento militare con il rango di Forza armata, ivi inclusa la sua partecipazione alle missioni internazionali. Nel dare risposta a questa interrogazione mi avvarrò prevalentemente di elementi forniti dal Ministero dell'interno, perché la tematica presentata è in gran parte attinente alle competenze di quest'ultimo Ministero. Sebbene l'eventualità di procedere alla soppressione della stazione carabinieri di Clodig (frazione del Comune di Grimacco) sia stata effettivamente presa in considerazione, dato anche il limitato impegno operativo (nel 2010 è stato perseguito un solo reato), il Comando generale dell'Arma dei carabinieri interessato la Legione carabinieri Friuli-Venezia Giulia per valutare la fattibilità e l'opportunità della modifica ordinativa - non ha adottato, ad oggi, alcun provvedimento al riguardo, né ha avviato l'*iter* procedurale per la richiesta del prescritto assenso da parte del Ministro della difesa, anche alla luce dell'auspicio espresso dal prefetto di Udine affinché il presidio possa continuare ad operare. In particolare, come immagino sia noto agli interroganti, la stazione ha competenza territoriale sui Comuni di Grimacco e Drenchia che si distinguono, peraltro, per le ottime condizioni di ordine e di sicurezza pubblica. Attualmente la stazione è ubicata in un immobile di proprietà dell'amministrazione comunale costruito nel 1960 e per il quale viene corrisposto un canone locativo annuo di 12.272 euro;

stabile. Qualora si dovesse procedere alla soppressione del reparto, ciò comporterebbe l'attribuzione del suo territorio alla giurisdizione della vicina stazione dei carabinieri di San Leonardo (distante circa 8 km), con la realizzazione di un dispositivo territoriale maggiormente rispondente

e alla tutela dell'ordine pubblico nell'area interessata, che sono stati sollevati dagli onorevoli interroganti. Ciò, nella consapevolezza che l'Arma dei carabinieri rappresenta una delle istituzioni più vicine ai cittadini, nei confronti dei quali svolge una costante azione di prevenzione quale espressione significativa della presenza dello Stato sul territorio.

è ancora un fronte abbastanza fragile rispetto ai passaggi e alle immigrazioni irregolari è importante. Presidi come questo, infatti, garantiscono, se non altro, una sicurezza e una rassicurazione che vanno confermate.

un seppur minimo Corpo di polizia municipale, laddove la presenza del comando dei carabinieri supplisce anche ai servizi che la polizia municipale può erogare sul territorio.

la prontezza e la compiutezza della risposta, ma non posso considerarmi del tutto rassicurato dalle prospettive che

Il sistema d'arma comunemente noto come *Joint Strike Fighter* (caccia F35, nella denominazione statunitense) è un programma pluriennale - la cui durata prevista è di circa quarant'anni - estremamente complesso e che prevede un forte coinvolgimento industriale, oltre ad essere di assoluto rilievo sia dal punto di vista strategico-militare che da quello operativo per le nostre Forze armate. L'Aeronautica militare e la Marina si doteranno di questo velivolo, che è idoneo ad assolvere le diverse missioni assegnate alle Forze armate italiane, anche in seno alle coalizioni internazionali. Come è noto, il velivolo sostituirà gli attuali velivoli AV-8B della Marina e gli AM-X e i Tornado dell'Aeronautica militare con un'unica linea, consentendo un incremento dell'efficacia operativa e una contestuale riduzione dei costi di supporto. Il JSF costituisce, dunque, la soluzione ottimale per il mantenimento di capacità essenziali nell'ambito degli obiettivi strategici posti alle nostre Forze armate, nonché perfettamente integrabile sia in contesti interforze, sia in quelli multinazionali, che sono tipici delle azioni fuori area. La partecipazione dell'industria nazionale al programma JSF si basa su piani di cooperazione - anche questi estremamente complessi - che al momento coinvolgono, per le fasi di sviluppo e di produzione, circa 30 aziende nazionali e prevedono un volume complessivo di opportunità per la nostra industria pari a circa 11,2 miliardi di dollari con l'azienda Lockheed Martin, a 2,4 miliardi di dollari con l'azienda motoristica Pratt & Whitney

i due gruppi è legata al fatto che sono attualmente in sviluppo due motori, tra i quali poi gli acquirenti potranno scegliere quello con cui equipaggiare il proprio velivolo. Riguardo alle ricadute in termini occupazionali, secondo una stima fornita dall'industria, la partecipazione al programma dovrebbe quantificarsi complessivamente in circa 10.000 posti di lavoro, mentre la struttura FACO/MRO&U (*Final Assembly and Check Out/Maintenance, Repair, Overhaul&Upgrade*), cioè la linea di montaggio finale, consentirebbe la creazione di circa 600 ulteriori posti di lavoro nella fase produttiva di picco, includendo in particolare manodopera altamente qualificata. Altre ricadute industriali, che sono ancora in corso di individuazione, potranno scaturire sia dalla fase successiva di sostegno logistico che dall'incremento della produzione legato alla vendita del JSF a Paesi che attualmente non fanno parte della *partnership* che produce il velivolo,

velivoli in un arco di circa trent'anni. In tale quadro, è stata fortemente sostenuta la scelta della realizzazione della linea finale di assemblaggio presso la base aerea di Cameri, in quanto soluzione da inserire in un sistema di supporto globale per svolgere attività successiva di manutenzione, revisione, riparazione e modifica di tutti i velivoli operanti nell'area europea e in quella mediterranea. La stessa capacità *FACO*, ovvero della linea di assemblaggio finale, rappresenta un'alternativa a basso costo e soprattutto a basso rischio, che potrà essere offerta per assorbire eventuali richieste produttive in eccesso rispetto alla capacità statunitense. La scelta della località è stata determinata sia dalla richiesta del Governo statunitense di realizzare, per ragioni di sicurezza, la linea di assemblaggio finale e di verifica, sia in base a criteri di competenza tecnica e di ottimizzazione delle risorse. Faccio presente che, come noto, nella citata area opera già il 1° reparto manutenzione velivoli dell'Aeronautica militare, che si occupa dei velivoli Tornado ed *Eurofighter*, e sono quindi presenti indubbie e pregiatissime competenze nel settore di interesse. Rispetto al tema della produzione delle ali a Cameri, faccio presente che in realtà si tratta di lavorazioni industriali che non concernono in termine tecnico la produzione stessa: essa viene infatti realizzata in stabilimenti dell'azienda italiana che si occupa di questo - la Alenia Aeronautica - in stabilimenti situati fuori dal Piemonte. Presso Cameri sarà invece effettuato l'assemblaggio delle componenti dell'ala: di fatto si parla dell'assemblaggio dell'ala e non della produzione delle singole componenti. In questo contesto risulta che, nel corso delle negoziazioni contrattuali, la Alenia Aeronautica ha concordato con l'azienda Lockheed Martin, capo-commessa della produzione dei velivoli,

Sottolineo che le scelte sulla località nella quale assemblare le ali del velivolo sono dettate da logiche di tipo industriale, rispetto alle quali il Ministero della difesa ovviamente non è intervenuto, se non prendendo atto delle determinazioni dell'azienda, che è - lo ripeto - la Alenia Aeronautica, responsabile della fornitura in questione.

l'ingegner Guarguaglini, presidente di Finmeccanica: sicuramente l'Alenia di Torino vivrà se sarà rifinanziata la terza *tranche* degli *Eurofighter*. Se non sarà rifinanziata, l'Alenia di Torino non vivrà. L'Alenia vivrà se il veicolo Vehicle*) potrà uscire dalla fase attuale, minima e sperimentale, realizzata prevalentemente con i fondi della Regione Piemonte, che speriamo siano riconfermati, anche se la produzione di questo velivolo è resa più difficile dagli ultimi accordi franco-britannici. Ciò che sta avvenendo nel polo aeronautico militare torinese e piemontese, è denso di grandissime implicazioni, l'una correlata all'altra. Per ciò che riguarda il senso del programma JSF, va tutto bene,

Riguardo ai soggetti citati nell'interrogazione, di cui all'articolo 12, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge n. 441 del 1982,

circa 800 dichiarazioni l'anno contenenti i dati sulla situazione patrimoniale e reddituale di chi ricopre cariche direttive di istituti ed enti pubblici; Relativamente poi ai casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri sia dovuto ricorrere alla diffida prevista dall'articolo 14 della citata legge nei confronti dei soggetti inadempienti, si fa presente che il Presidente del Consiglio dei ministri non è mai ricorso alla diffida. invece dato luogo ad apposite circolari, direttive e solleciti, rivolti a tutti i Ministeri e da enti interessati, con cui è stata richiamata l'attenzione sugli adempimenti previsti dagli articoli 12 e seguenti della suddetta legge n. e sull'obbligo, per i titolari di cariche direttive di istituti e di enti pubblici, di inoltrare ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione relativa alla propria situazione reddituale e patrimoniale

Per quanto concerne la pubblicità data alle dichiarazioni dei soggetti di cui al suddetto articolo 12, i dati raccolti sono pubblicati in appositi bollettini annuali redatti a cura del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, sia in forma cartacea che in forma elettronica, Questi bollettini, oltre ad essere inviati alle varie amministrazioni dello Stato e a tutte le prefetture, sono disponibili per la consultazione, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Della pubblicazione dei bollettini e delle modalità di consultazione viene annualmente data notizia attraverso un apposito comunicato stampa. Inoltre, ogni anno, in occasione del Forum della pubblica amministrazione, gli stessi bollettini sono presenti negli *stand* del Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Sottolineo, infine, che il bollettino per l'anno 2010 è stato pubblicato il 29 aprile 2011. ringrazio il sottosegretario Cossiga per la risposta, estremamente puntuale.